preso atto, almeno qui dentro, di un fatto cruciale e cioè un cambio di maggioranza, giacché nei successivi voti di fiducia che si sono inanellati come una triste litania abbiamo visto entrare in maggioranza un Gruppo parlamentare e uscirne un altro. Sono cambiate le architetture

alle prescrizioni della legge di contabilità. Bene, in questo momento cruciale per tante famiglie e imprese noi assistiamo ad un cambio di maggioranza che, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere immediatamente formalizzato al Presidente della Repubblica.

come Capogruppo, può fare le dichiarazioni sull'ordine dei lavori, però andiamo avanti, come richiesto da lei stesso, con le dichiarazioni di voto in diretta televisiva. Dopodiché avrà tutta la possibilità di parlare.

legge sui partiti, con riferimento alla democrazia interna, ai codici etici, all'accesso alle candidature e al finanziamento, e la legge elettorale con il doppio turno. Nulla di tutto ciò è avvenuto. Dopo cinque anni di fallimenti istituzionali e democratici, in quest'Aula la democrazia interna dei partiti non esiste; anzi, è osteggiata con pratiche e manovre indicibili. Ciò che state per approvare è palesemente incostituzionale, anche questa volta. L'unico scopo è il mantenimento dello *status quo* delle vostre organizzazioni inginocchiate alla volontà di pochi. La proposta del PD è rinnegata dai fatti nei suoi propositi. Per molti sarà motivo di rimpianto, di rimorso e per altri di rimborso. Consolatevi. *Senatores boni viri, Senatus mala bestia*. Secondo l'articolo 48 della Costituzione: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». L'esercizio di quel voto, che ora attuerete stravolgendolo, non è eguale perché non è uguale il destino di quel voto se è dato in contesti differenti e non è libero, e dunque non democratico, perché quattro capi di partito diranno a tutti chi votare. Legge elettorale *erga omnes*?

Concludo dicendo che la governabilità è certa solo nella monarchia, nella democrazia non è data dalla legge elettorale ma esclusivamente dalla capacità politica di convergere, con mediazione, dialogo e confronto, verso i bisogni di un Paese e non verso i vostri.

in questi giorni ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori, ma credo che con l'approvazione di questa legge elettorale oggi il Parlamento compia un atto di responsabilità verso il Paese. Non è una legge elettorale perfetta, ma dopo la vittoria del no al *referendum*, questo era l'unico accordo possibile con il più ampio consenso possibile. Discutere sulla fiducia o no è, dunque, pura ipocrisia perché, a pochi mesi dalla fine della legislatura, se si vuole davvero scongiurare il periodo di andare a votare con due sistemi diversi nelle due Camere, il che getterebbe il Paese nel *caos*, questo è ciò che si deve fare. Tutti sappiamo che con l'Italicum e la riforma costituzionale gli italiani avrebbero davvero potuto scegliere da chi essere governati, dando anche vita a un sistema di Governo più semplice e efficiente. È stato un errore enorme bocciare la riforma costituzionale, così come sappiamo che il sistema proporzionale nel quale ci stiamo avviando guarda - ahimè - più al passato che al futuro. Anche se, volendo dirla tutta e dovendo essere sinceri, certe coalizioni eterogenee, incoraggiate dai sistemi maggioritari e nate solo per vincere le elezioni, non hanno dato granché buona prova di governo. Dunque questa legge è la soluzione migliore per evitare il peggio e abbiamo il dovere di approvarla, mettendo da parte inutili polemiche. In fondo il futuro dell'Italia non lo si gioca con la legge elettorale: il futuro dell'Italia si gioca sui programmi delle forze politiche. Infine, signor Presidente, non temo l'eventuale formazione di Governi di unità nazionale nella prossima legislatura, un po' perché in tutta Europa ormai questa formula è all'ordine del giorno, un po' perché oggi la stessa frammentazione dell'opinione pubblica italiana, forse in questa particolare fase storica, chiede Governi di coalizione, che però mi auguro siano formati da forze convintamente europeiste per frenare la pericolosa ondata populista che oggi abbiamo in tutta Europa. Con questo spirito dichiaro di votare convintamente a favore del provvedimento. Signor Presidente, non ho partecipato ieri ai voti di fiducia, in quanto, considerando meritevole di fiducia il Governo Gentiloni Silveri, avrei dovuto votare sì, ma questo mi avrebbe portato a esprimere sostegno al disegno di legge al nostro esame che non condivido nel merito. In sede di voto finale, sul quale non è posta la questione di fiducia al Governo,

Mi limito a ricordare l'impossibilità del voto disgiunto, l'indicazione del nome del capo della forza politica

Napolitano - sono state imposte al Governo e, di fatto, ai singoli parlamentari temo non contribuiranno a dare ai cittadini il senso della serietà della politica. Temo invece che contribuiranno a diffondere il disprezzo nei confronti della politica. Signor Presidente, colleghi senatori, il giudizio su una legge elettorale non risponde né a esigenze etiche né tantomeno a tensioni di tipo ideale. La legge elettorale è uno strumento che serve innanzi tutto a tradurre i voti in seggi, garantendo nel contempo, e per il possibile, rappresentanza e governabilità. Per svolgere bene il suo compito, essa deve armonizzarsi con la situazione storica e il contesto istituzionale. Se non si accetta questa premessa non si comprende perché uomini come Luigi Sturzo e Gaetano Salvemini - che nel 1919 erano stati padri del proporzionalismo - all'alba della storia repubblicana, in un diverso contesto, si trovarono a prendere posizione per il sistema maggioritario. Se non si accetta questa premessa non si riesce a capire perché, quando il percorso delle riforme è partito, all'inizio di questa legislatura, si era pensato che la legge elettorale dovesse seguire la riforma delle istituzioni e non anticiparla. Solo così, infatti, si sarebbe potuto considerare l'assetto istituzionale nel quale la nuova legge si sarebbe collocata. Solo così si sarebbe potuto valutare se il superamento del bipolarismo sancito chiaramente dalle urne nel 2013 si fosse nel frattempo consolidato o se, al contrario, i due schieramenti storici - centrodestra e centrosinistra - fossero stati in grado di riassorbire il voto di protesta confluito sul Movimento 5 Stelle, Com'è noto, lo schema iniziale è saltato. Il precedente Governo ha imposto l'approvazione dell'Italicum, con l'intento di cambiare surrettiziamente la forma di Governo introducendo dalla finestra quel premierato che avrebbe dovuto entrare dalla porta principale assieme ai suoi contrappesi, e ristabilendo per legge elettorale un bipolarismo di fatto ancora più in crisi di quanto lo fosse nel 2013. Si potrebbe obiettare che Renzi non è stato certamente il primo in Italia ad aver assegnato alla legge elettorale compiti impropri. È vero, ma forse mai si era arrivati a forzare a tal punto la mano. Così, a valle di questa forzatura ci siamo trovati in un vero e proprio disastro: con due leggi elettorali scritte dalla Corte costituzionale e non dal Parlamento, compilate in tempi differenti e, come si sa, redatte procedendo per "sottrazione" delle loro parti incostituzionali al solo fine di evitare un vuoto normativo. Ne è venuto fuori, inevitabilmente, un prodotto segnato da assoluta incoerenza. Il Consultellum del Senato incoraggiava le coalizioni, quello della Camera non le contemplava; la legge del Senato non prevedeva premio di maggioranza, quella della Camera sì; per il Senato c'erano collegi grandissimi, per la Camera molto piccoli; il sistema del Senato apriva totalmente alle preferenze mentre quello della Camera, bloccando i capilista, avrebbe determinato un'Assemblea fatta in maggioranza da nominati; la legge del Senato non prevedeva voto di genere, quella della Camera sì; le due leggi, inoltre, dettavano regole differenti sugli sbarramenti e sulle multicandidature. Grazie, non possiamo fare a meno di considerare le macerie dalle quali proveniamo, e pensare per un attimo alla prospettiva alternativa che ci sarebbe stata imposta: quella di provare a mettere ordine, per il poco possibile, utilizzando uno strumento inopportuno come un decreto-legge varato all'ultimo minuto prima che l'arbitro fischi la fine della partita. Insomma, non possiamo non valutare cosa, in alternativa a questa legge, ci sarebbe potuto toccare in sorte. In quest'ottica, iniziamo col dire che alcuni elementi di questo disegno di legge non ci piacciono. Innanzi tutto - lo ribadiamo l'apposizione della fiducia, sostanzialmente sull'intera legge elettorale, è stata un atto improprio. È vero, presidente Napolitano, che questa inappropriatezza non è statuita da una sentenza della Corte costituzionale, ma le istituzioni vivono anche di consuetudini, e queste talvolta entrano nella sfera intangibile della *iurisdictio*, anche in sistemi regolati da norme scritte. E il fatto che le leggi elettorali debbano derivare da un libero dibattito parlamentare appartiene certamente alle consuetudini della nostra storia repubblicana. Avevamo apprezzato che il presidente Gentiloni Silveri, nel suo discorso di insediamento, avesse mostrato di voler recuperare questa usanza riparando a uno sbrego operato dal suo predecessore. Purtroppo è stato costretto a contraddirsi. Nel merito, non ci piace l'esiguità dello spazio riservato alla scelta dei cittadini. Lo dico anche contro gli interessi della mia parte politica, ma credo che questo spazio si sarebbe potuto ampliare prevedendo il voto disgiunto, e ciò avrebbe potuto valorizzare ancor di più la qualità delle persone chiamate a rappresentare i diversi schieramenti nei collegi uninominali. Ancora, non ci piace la norma sugli italiani all'estero. Avremmo voluto, sul punto, una riforma più radicale che rilanciasse il significato di quella rappresentanza. Non ci pare che consentire la candidatura oltreconfine ai residenti in Italia vada in questa direzione. Non ci convince del tutto, infine, la norma sulla parità di genere. Non perché prevedere un qualche meccanismo che bilanci una situazione di squilibrio determinata da ragioni storiche e sociali non sia legittimo. Ma perché tale normativa, per non assumere un significato impropriamente corporativo che finisce col danneggiare il merito di chi vorrebbe tutelare, deve essere immaginata come temporanea e tradursi in meccanismi più semplici di quelli che presiederanno la compilazione delle prossime liste elettorali. Va detto tuttavia - mi permetta una nota di leggerezza - che questa norma porta con sé una conseguenza che certamente non piacerà ai sostenitori della teoria *gender* e a quanti ritengono che la sessualità sia fluida e possa essere determinata da fattori solo culturali. Il voto di genere riafferma infatti l'identità sessuale, giacché per poter partecipare a una competizione devi sapere chi sei. Quanto meno al momento di candidarti! Su un altro versante, la legge che ci accingiamo a votare presenta però degli indubbi vantaggi. Innanzitutto incoraggia le coalizioni, che non sono certamente il "bene assoluto", ma in questo momento storico rappresentano la soluzione che più può avvicinarci all'obiettivo di dare al nostro Paese un Governo stabile. nella selezione delle candidature, e a minoranze creative e raggruppamenti civici di essere rappresentati nel prossimo Parlamento. Infine

limitando la regionalizzazione della rappresentanza nella Camera alta alla sola ripartizione dei resti. In tal modo - va da sé - sarà molto più probabile avere nei due rami dell'assemblea maggioranze omogenee. C'è tuttavia un aspetto che va al di là di tutto ciò. In un Paese civile, infatti, le leggi elettorali le scrivono i Parlamenti, non i giudici. In Italia, inoltre, i giudici costituzionali autori del Consultellum e del Consultellum 2 non ambivano ad arrogarsi la scrittura di quelle norme, e nell'ultima sentenza avevano lanciato un ammonimento che nella sostanza suona così: «Noi non siamo legislatori e non possiamo produrre diritto positivo. Per evitare vuoti normativi abbiamo dovuto recuperare persino istituti bizzarri come quello del sorteggio. Cari parlamentari, tocca a voi scrivere la riforma. Anche perché i prodotti dei nostri due pronunciamenti, considerati insieme, possono presentare tratti di incoerenza così evidenti da risultare incostituzionali». Chi ha letto l'ultima sentenza della Corte sa, sa, insomma, che essa conteneva un messaggio in bottiglia per il Parlamento e per la politica. Non tutti gli aspetti del provvedimento oggi al nostro esame sono certamente esenti da censura, ma quantomeno ci si è tirati fuori da una situazione di illegittimità acclarata. Se il Parlamento non fosse intervenuto - come in alcuni momenti abbiamo temuto - questa inerzia avrebbe inferto una ferita ancora più profonda alle istituzioni e accertato la paralisi della politica e dei partiti. in questi giorni, in questo emiciclo è stata data una prova di vitalità, anche e persino attraverso le proteste irrituali di alcune delle forze che si oppongono a questo Senza dubbio, meglio tutto ciò che la morta gora. Ed è per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo Federazione della Libertà. *(Applausi Signor Presidente, intervengo questa mattina perché nel dibattito sulla riforma elettorale sono stato "tirato per la giacca", da chi mi ha evocato e da chi mi ha insultato. A chi mi insulta non rispondo, perché voglio parlare solo ed esclusivamente di politica. Dovrei dire «*ecce homo*», con tutto quello che ho ascoltato. Credo sia giusto e opportuno essere qui Credo sia giusto e opportuno essere qui per rispondere, spiegare e chiarire. Prima di tutto voglio dire che, a mio parere, questa è una buona legge elettorale; non è un colpo di mano, tantomeno un colpo di Stato. Le parole in politica sono pietre e dovrebbero essere soppesate prima di gettarle nelle arene popolari. Ovvio, non è la migliore legge elettorale, perché leggi perfette in questo ramo del Parlamento e nell'altro non esistono. Ma è la migliore possibile in questo momento storico e in questo Parlamento.

Dicono che la legge sia figlia mia, il che non mi dispiace, però direi che forse è nipote, perché era un'idea che è stata poi sviluppata. È una legge necessariamente frutto di un compromesso, ma onestà intellettuale vorrebbe che si aggiungesse a ciò che tutta questa legislatura è stata un compromesso, un grande compromesso. Troppo spesso si finge di dimenticare il risultato del 2013: elezioni che non produssero una maggioranza politica. Le alternative erano: o sciogliere le Camere o cercare un punto d'incontro tra le forze politiche responsabili. Ebbene, c'è stato e oggi si dice che si è realizzata una maggioranza con l'uscita di Articolo 1 - MDP e con il nostro ingresso. Non è vero. Non è vero, perché noi c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo fino all'ultimo giorno della legislatura.

Nel silenzio, ci è sempre risultato incomprensibile questo atteggiamento sofistico dei pitagorici di quest'Assemblea, i quali sono specializzati nella semplice aritmetica e non hanno mai compreso la politica; o forse hanno fatto finta di non comprenderla. La nostra scomoda presenza ha sterilizzato i massimalismi *post-*comunisti e gli integralismi cattolici, che vivono ancora con la testa nel passato e i piedi nel trapassato,

e tutto quello che è stato detto nei nostri e nei miei confronti li valuto soltanto come atti politici. Come ho detto, non rispondo alle offese, perché al di là dei retaggi e delle nostalgie, in fondo, per la storia, la sinistra rispetto alle idee si confronta anche in modo polemico e in modo forte. Capisco l'amarezza dei cosiddetti bersaniani (verdiniani, bersaniani...).

In quest'Aula, quando si è trattato di contare i nostri voti, si è rinnegata persino l'aritmetica (a qualcuno regalerò un abaco). Ma questo consente di rivendicare con orgoglio a me stesso e al mio Gruppo tutto quello che abbiamo fatto, a partire dal ruolo di supplenza politica che abbiamo svolto, tutelando la stabilità e l'interesse del Paese. Ogni volta che un provvedimento ci è sembrato giusto e andare nella giusta direzione lo abbiamo sostenuto, ignorando gli stupidi strali che ci venivano quotidianamente rivolti. Noi siamo quelli che hanno consentito al Paese di fare uno scatto in avanti sul fronte dei diritti, rendendo possibili le unioni civili, e avremmo votato anche la *stepchild adoption*, così come voteremo il testamento biologico, quando e se arriverà in Siamo quelli che hanno contribuito a mettere in sicurezza i conti pubblici, votando i DEF senza essere in maggioranza, "Ministri senza portafoglio". E poi siamo stati leali con Letta, con Renzi e anche con Gentiloni Silveri, nonostante la sua costante indifferenza. Signor Presidente, vengo a un argomento per me indubbiamente scomodo. ho problemi giudiziari. Ho sempre rispettato i giudici e la giustizia. Mi sono difeso nei processi e non dai processi e pretendo, come tutti, il rispetto costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Ma in quest'Aula, stranamente, la grande difesa della bellissima Costituzione talvolta si dimentica e si approfitta strumentalmente delle mie questioni giudiziarie, che nulla hanno a che spartire con la mia e con la nostra azione politica, rendendo inefficace la fattiva presenza in Parlamento, che è stata costantemente derubricata, osteggiata e vilipesa. Un tempo, esisteva l'appoggio esterno ai Governi. Adesso c'è l'appoggio fantasma: un neologismo tartufesco appositamente per noi, perché sanno anche i sassi che qui dentro non c'è mai stata una vera maggioranza politica con la quale tutti devono fare i conti.

Tutti, fra deputati e senatori che hanno cambiato Gruppo, sono traditori o è l'effetto dei mutamenti politici e della stagione politica? Perfino gli amici di Articolo 1 hanno cambiato maglia, Fucksia).* Anzi, noi siamo stati il grillo parlante del riformismo, aiutando spesso il PD a compiere scelte difficili, mettendo a nudo le contraddizioni fra le sue due anime, sull'innovazione costituzionale, sulle politiche del lavoro, sul *jobs act*, con l'abolizione dell'articolo 18, sull'IMU prima casa - un bene inestimabile per tutti, poveri e ricchi sull'IRAP, sul superammortamento e sulla rottamazione delle cartelle. Quando sosteniamo questo, ci chiamano renziani. Abbiamo dato fastidio a tutti e qualcuno ha tentato di schiacciarci non c'è riuscito, ma forse perché abbiamo capito la nuova fase politica prima di altri e lo vedremo. Fa scandalo affermare che non ci sono più destra e sinistra e - per dire la verità - suona strano anche a me. Ma è difficile negare che oggi la sfida delle democrazie occidentali sia non più fra destra e sinistra, ma fra apertura alla modernità e chiusura nel passato. E lo dimostra questa drammatica legislatura: abbiamo eletto due Presidenti, abbiamo votato tre Governi, varato due leggi elettorali, l'antipolitica ha gonfiato le vele, Berlusconi è stato espulso infaustamente da questo Senato, il patto del Nazareno è fallito, la riforma costituzionale è stata bocciata; una navigazione davvero difficile per tutti. Berlusconi, che ho ricordato, è stato il grande innovatore della politica e la storia glielo riconoscerà, ma mi pare che in questi tempi lo riconosca anche sua lotta riformista, credendo e sperando poi nella forza innovativa di Renzi, per portare a conclusione l'indispensabile trasformazione e transizione del Paese. Ma, se anche il patto del Nazareno è imploso, noi abbiamo continuato a lavorare e a credere nell'unione delle forze migliori del Paese, per ostacolare le derive i cui esempi si possono leggere in tutta Europa e in tutto il mondo. È una necessità storica, determinata dalla globalizzazione, dalla crisi economica, dalle migrazioni impetuose: un fenomeno che è illusorio voler fermare alzando muri, ma che va governato con politiche di sicurezza e di integrazione e con una grande coesione nazionale. Per quel che mi riguarda, ma lo dico a titolo strettamente personale, io sarei pronto a votare lo *ius soli*, anche domani, in coerenza con quanto già fatto per la legge sui minori non accompagnati. Sono costretto, Presidente, a chiudere questo intervento - annunciando il mio voto favorevole - facendo riferimento ancora una volta alla mia persona. Con questa riforma viene consentito di candidarsi all'estero una delle tante, stupide, falsità dette sul mio conto. Io non so se mi ricandiderò ma, se lo farò, lo farò sicuramente in Italia. Se mai un giorno, e non lo auspico, il Veneto e la Lombardia conquistassero l'indipendenza, forse potrei candidarmi là, per battermi, da vecchio repubblicano, per l'unità del Paese.

La materia elettorale è da prendere con le pinze - come si suol dire - e, anche se forse ingiustamente, mi viene attribuita una certa conoscenza della materia, conoscenza che deriva dal fatto che, diversamente da altri, io ho provato il sistema proporzionale con le preferenze; ho provato il cosiddetto Mattarellum e ho provato il cosiddetto Porcellum. E oggi vi posso dire con tranquillità che, in un sistema tripolare come quello attuale, non esiste e non può esistere una legge elettorale perfetta. Questo ve lo dico chiaro e tondo. Parlo di conoscenza della materia perché, prima

ho fatto i nomi e i cognomi dei responsabili che hanno rovinato quella legge e nessuno ha mai smentito. Sono stato ingiusto a definirla una porcata. Non userei più quel termine, perché le porcate sono venute dopo, con la responsabilità di tanti seduti in questo Parlamento. Porcata era una riforma costituzionale che instaurava un regime di monarchia. Porcata era una legge elettorale, l'Italicum, pensata per il signor Renzi solo al comando. Porcate sono quattro Presidenti del Consiglio mai eletti da nessuno e sostenuti da persone elette nel centrodestra

La Corte costituzionale ha detto che doveva essere completata con atti normativi di rango primario o secondario. Eravamo nel gennaio 2014. Da allora nessuno ha fatto niente. Se si fossero sciolte le Camere, non ci sarebbe stata la possibilità di tornare al voto, oppure si tornava al voto con un decreto ministeriale impugnabile davanti a un qualunque TAR. Quella situazione non avrebbe consentito l'esercizio della democrazia: se un Paese non può votare, è stata sospesa la democrazia.

a cena o a pranzo, se devo scegliere un vino, prendo quello bianco o quello rosso; il rosatello non l'ho mai preso in vita mia. Piuttosto che l'acqua, però, prendo anche il rosatello.

avrei scelto il Mattarellum, con due terzi maggioritario e un terzo proporzionale, o un premio di maggioranza per garantire un po' di più quella governabilità,

Lo dico con sincerità ai nostri compagni della maggioranza. Ragazzi miei, *l'è finida*. Siamo alla frutta, anzi è arrivato addirittura il conto, ormai: ve lo presenterà il popolo quando tornerà a votare.

piaccia o no. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Mi scuso con il collega Razzi, perché userò una sua espressione. "Ve lo dico da amico": fermate il pazzo. Ragazzi miei, nei mille giorni di Governo ha distrutto il Paese

approvare una legge elettorale che probabilmente determinerà l'estinzione del suo partito. È diventato imbarazzante! Adesso si è messo anche a giocare col treno. Ragazzi, tenetelo sul treno perché, se scende, qualcuno lo aggredisce. Un tempo giocava alla playstation con Orfini. Comprategli un bel plastico e fatelo giocare con la Boschi, con Orfini e col "giglio magico", ma fermatelo, perché è pericoloso per sé e per gli altri.

A chi disturba gli interventi degli altri voglio ricordare una cosa. Avete parlato di attentato alla democrazia, avete rifiutato la fiducia, e avete fatto bene. Io ero invidioso quando avete occupato i banchi del Governo. Ma, dopo averlo fatto, sarei rimasto lì tutta la notte e non mi sarei mai mosso. Non è giusto, dopo aver parlato di attacchi alla democrazia e tutto il resto,

Se la democrazia può essere svenduta per una diretta televisiva, ragazzi miei, voi fate parte della commedia, ma alle prossime elezioni sarete solo delle comparse.

riconoscendo e rispettando le ragioni di altre componenti dello stesso Gruppo che vorranno esprimere una scelta opposta. Se siamo arrivati solo oggi a votare la nuova legge elettorale, a pochi mesi dalla scadenza naturale di questo Parlamento; se abbiamo dovuto fare una rincorsa per arrivare a un testo incompleto - con i difetti prima segnalati - e non decisivo per il nuovo Parlamento, l'unico responsabile è il segretario del Partito Democratico. Qualora dovessimo avere dei vuoti di memoria, basterà andare a rileggere la gran parte degli interventi formulati nella discussione generale sull'Italicum. In essi, oltre a censurare nel merito la legge e l'opportunità del sistema elettorale prescelto, si evidenziavano i gravi vizi di incostituzionalità del testo normativo. Ma, anche in quel caso, così come in quello più eclatante della riforma costituzionale, l'arroganza e la stupida pervicacia dell'allora *Premier* prevalsero, imponendo al nostro Paese una legge che, due anni dopo, è stata dimezzata dalla sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale. In questi giorni, chi ha osteggiato il presente disegno di legge ed è stato escluso dall'accordo sul cosiddetto Rosatellum ha evidenziato che l'approvazione della legge sul finire della legislatura si pone in contrasto con il paragrafo 65 del Codice di buona condotta in materia elettorale del Consiglio d'Europa. Tutti abbiamo letto si dice che: «Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito». se si è arrivati a violare anche questa disposizione, la responsabilità politica è sempre quella del PD e del suo segretario, che hanno tenuto in scacco per tre anni l'intero Parlamento nella prospettiva di una consistente modifica della Costituzione, che - più che una riforma - era un falso tentativo di cambiare la Carta, sgrammaticato e lontano anni luce da quanto chiedevano gli italiani. Il 4 dicembre gli elettori hanno, infatti, bocciato tale perverso disegno e, tra gli effetti di quel no al *referendum*, ci è rimasto un Italicum falcidiato dalla Corte, peraltro utilizzabile solo per l'elezione della Camera dei deputati. Quindi, tre anni di discussioni inutili hanno determinato questo *forcing* sulla legge elettorale, costringendo le Camere ad approvarla in pochissime settimane. Ciò nonostante, questo Parlamento ha il dovere di risolvere l'attuale *impasse* sul sistema elettorale. Se non approvassimo oggi un nuovo testo, costringeremmo gli italiani ad andare al voto con il sistema vigente. L'elezione del Senato sarebbe regolata dalle previsioni della legge Calderoli del 2005, così come rimaneggiata dalla Corte nel gennaio del 2014. Utilizzeremmo, in tal modo, un sistema proporzionale puro, basato su un collegio unico regionale con voto di preferenza, che vedrebbe eletto solo il *leader* di un partito, o un suo preposto, o un candidato plurimilionario molto facoltoso o, ancor peggio, sostenuto da organizzazioni criminali. Alla Camera dei deputati, poi, si dovrebbe ricorrere al cosiddetto Italicum costituzionalizzato, nel quale è sopravvissuta la soglia del 40 per cento per ottenere il premio di maggioranza. Come si vede, se si votasse oggi con un sistema elettorale altamente disomogeneo, si avrebbe la possibilità di una maggioranza piena solo alla Camera dei deputati, con un Senato balcanizzato e non governabile. Di fronte a questo quadro disomogeneo, nella scorsa primavera il Partito Democratico ha fatto la proposta scabrosa del cosiddetto Tedeschellum, che aveva solo il pregio di un'apparente larga condivisione parlamentare, ma nel contempo evidenziava larghi difetti, tra i quali la fragilità dello stesso accordo - infrantosi su uno dei primi voti segreti - e l'impossibilità matematica di far conseguire a qualsiasi partito una maggioranza parlamentare. Attraverso questo percorso accidentato siamo giunti all'attuale disegno di legge, non cito il nome, non riconoscendo al proponente alcuna particolare competenza tecnica o abilità scientifica. Alcune novità del testo sottoposto alla nostra approvazione sono certamente apprezzabili.

Siffatta previsione del disegno di legge induce a optare per un voto favorevole, ma molti restano i vizi che in un dibattito parlamentare meno coartato e non contingentato avremmo voluto eliminare o ridurre. Certamente sarebbe stato auspicabile un numero maggiore di collegi uninominali, magari tornando alla misura prevista dal cosiddetto Mattarellum (75 per cento) o, almeno, a una divisione paritaria con gli eletti nel plurinominale proporzionale. A tal fine, avevo proposto degli emendamenti, purtroppo preclusi dalla scelta del voto di fiducia di ieri. Inoltre, non è soddisfacente l'eccessiva estensione territoriale dei collegi della quota proporzionale. Il rischio, in questo caso, è è quello della scarsa conoscenza del candidato, così come aveva già indicato la Consulta nella sentenza n. 1 del 2014. Il difetto maggiore è, comunque, quello prima evidenziato, della ridotta quota di maggioritario, che non potrà determinare in modo significativo l'esito della competizione elettorale. Altra questione dibattuta che lascia perplessi è quella del meccanismo dell'unico voto per il collegio maggioritario e per quello proporzionale. Una maggiore meditazione avrebbe potuto condurre a riflettere sull'opportunità di siffatta previsione, evitando i sicuri strascichi di una futura *querelle* dinanzi alla Corte costituzionale. Pur tuttavia, le evidenziate ragioni riguardanti la necessaria eliminazione del vigente sistema elettorale, disomogeneo e per nulla organico, mi inducono a una valutazione complessivamente favorevole del presente disegno di legge. Resta l'amarezza per quello che si poteva fare in questa legislatura e non si è fatto. Aumenta il rimpianto per la mancata riforma del nostro assetto costituzionale, dissoltasi per la vanagloria del segretario del PD, che da Presidente del Consiglio ha venduto l'illusione di un sistema istituzionale fondato sulla certezza di un vincitore delle elezioni e di una granitica maggioranza parlamentare. Così non è stato. Nessuno, a cominciare dal segretario del PD, ha fatto i conti con lo scenario attuale, come ricordato prima dal collega Calderoli: mi riferisco a un sistema politico tripolare, che che determina, sulla base di leggi elettorali proporzionali, una stagione perenne di Governi di larghe intese, ovvero situazioni perduranti di *impasse* parlamentare. Come si sarebbe potuto evitare questo rischio? Certamente non con la proposizione di modelli basati su consistenti premi di maggioranza, come avviene per le elezioni regionali. In quel caso, il rischio sarebbe una nuova pronuncia di incostituzionalità, come avvenuto per la legge del Forse l'unica via, suggerita da noi e da molti altri esponenti del centrodestra durante la gestazione delle riforme costituzionali, sarebbe potuta essere quella dell'evoluzione del nostro sistema costituzionale verso la forma del presidenzialismo, cui avrebbe fatto da corollario una legge elettorale a doppio turno, unico antidoto alla paralisi dell'Italia tripolare. Ciò non è avvenuto perché si è pensato agli effetti taumaturgici della riforma Boschi e dell'Italicum, che avrebbero garantito - così si diceva - la piena governabilità del nostro Parlamento. gli elettori, il 4 dicembre, non hanno avuto la stessa opinione e oggi, con questa legge, cerchiamo di ridurre il danno di una pessima stagione di Governi a guida PD, già ripudiati dagli italiani e ormai da collocare nel dimenticatoio. Proprio per quest'ultimo motivo e per conseguire l'obiettivo di risolvere l'attuale paralisi del nostro sistema elettorale, confermo il voto favorevole annunciato all'inizio del mio intervento.

forse non ottimale, ma sicuramente realistico, nel quadro difficile e complesso determinato dalla rottura del patto politico, che nel giugno di quest'anno era stata prodotta in Aula alla Camera, nonostante il cosiddetto Tedescum fosse stato già votato in Commissione dalle forze politiche rappresentative di ben l'80 per cento In tempi normali, anche noi saremmo stati contrari ad approvare la legge elettorale a colpi di fiducia, e in questo senso condividiamo le perplessità espresse dal presidente Napolitano, ma i tempi non sono normali. È l'ultima occasione per questo Parlamento per dimostrare di essere in grado di fare una legge elettorale e di garantire regole certe per le prossime - e ormai non troppo lontane - elezioni. Il presente testo uniforma i sistemi elettorali di Camera e Senato ed è appoggiato dalla maggioranza e anche dalle opposizioni, come auspicato dal presidente Mattarella, e questo è positivo. Consentitemi però anche di muovere una considerazione nella mia veste di esponente delle minoranze linguistiche. Negli ultimi giorni sono stato oggetto di pesanti critiche, anche sul piano personale,

come già avvenuto nel corso delle votazioni sulla riforma costituzionale - di utilizzare le norme regolamentari, che consentono il voto segreto per le questioni riguardanti le minoranze linguistiche, per fini del tutto estranei alle minoranze stesse e certamente non nel loro interesse. Anzi, gli emendamenti del Movimento 5 Stelle non hanno nulla a che fare con la tutela delle minoranze linguistiche. *(Commenti dei

e di garanzia previste dalla Costituzione. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti a prima firma Endrizzi, Morra e Crimi, tutti senatori del Gruppo Movimento Caro senatore Endrizzi, non è per nulla convincente il modo con cui due giorni fa in quest'Aula ha cercato di giustificarsi. I suoi emendamenti parlano chiaro: sono non solo incostituzionali, ma addirittura fortemente discriminatori nei confronti delle minoranze linguistiche, e vi spiego subito il perché.

e i voti per i candidati nei collegi uninominali sia per la Camera che per la legge elettorale in discussione non prevede più lo scorporo e i voti per i candidati nei collegi uninominali sia per la Camera che per il Senato vengono conteggiati anche per l'assegnazione dei seggi per la parte proporzionale. Cosa proponeva però il Movimento 5 Stelle? LUCIDI *(M5S)*. Stelle proponeva che, per le sole minoranze linguistiche, venisse applicato un sistema di scorporo estremamente penalizzante e discriminatorio, togliendo tutti i voti dei candidati nei collegi uninominali per il sistema proporzionale e ciò solo per le minoranze. I voti per il Movimento 5 Stelle valevano al 100 per 100, quelli per le minoranze non dovevano valere nemmeno la metà. Questo è davvero sconcertante

Non so perché il Movimento 5 Stelle crede che i partiti espressione delle minoranze linguistiche non debbano poter concorrere per l'assegnazione dei cinque seggi nel Trentino Alto-Adige Südtirol, previsti per il proporzionale. Non lo so.

Avrei difeso un sistema elettorale che garantirebbe sette seggi per la Regione Trentino Alto-adige Südtirol,

Caro collega Marton, capisco che nella sua vita precedente aveva poco a che fare con sistemi elettorali. *(Commenti dal Gruppo M5S).* Credo però che un cittadino medio, ma soprattutto un senatore della Repubblica, dovrebbe almeno conoscere la Costituzione italiana. Vada a leggersi, per esempio, il comma 3 dell'articolo 57. Anzi, glielo leggo io: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette», per cui anche la Basilicata con 700.000 abitanti ha sette senatori e chiaramente anche la Regione Trentino con un milione ha sette senatori. Dove starebbe, quindi, il privilegio del Trentino-Alto Adige Südtirol? La prossima volta, prima di prendere la parola in quest'Aula, dovrebbe leggere la Costituzione!

in questa Assemblea. Il che corrisponde alla nostra forza politica sul territorio e ai voti dati dai nostri cittadini. In base a cosa continuate a dire che la SVP alle prossime elezioni farà sette senatori su sette? È proprio una critica assurda.

ma anche per noi e, d'altra parte, non siete stati voi stessi a far saltare l'accordo del giugno scorso, chiedendo di estendere

Quindi, non lamentatevi ora che il Parlamento ha fatto esattamente quello che chiedevate con gli identici emendamenti di Fraccaro e Biancofiore. Abbiamo esteso il sistema di voto vigente per tutta Italia anche a Bolzano per i seggi proporzionali. Cosa volete, allora?

come Autonomie e minoranze linguistiche intendiamo, comunque, ribadire le ragioni costituzionali e statutarie per le quali per il Trentino-Alto Adige Südtirol sono stati confermati i sei collegi uninominali per Camera e Senato. Come sappiamo, i sei collegi uninominali al Senato, di cui tre nella Provincia autonoma di Bolzano, sono frutto di un accordo internazionale e derivano dal cosiddetto Pacchetto del del 1969 fatto con l'Austria e sono, per tale ragione, sopravvissuti come *unicum* in tutta Italia anche al Porcellum del 2005 - per questo sono stato eletto con il Mattarellum - che aveva abolito (come è noto) il sistema dei collegi uninominali in tutta Italia, ma non per il Senato nostra Regione. Stante l'esigenza di uniformare il sistema di voto di Camera e Senato e per favorire la rappresentanza di tutti i Gruppi linguistici presenti sul territorio, il sistema elettorale con tre collegi uninominali nella Provincia di Bolzano, già in vigore per il Senato, è stato giustamente esteso anche alla Camera. Il sistema ha, inoltre, il grande pregio di garantire la presenza delle minoranze linguistiche a prescindere dal superamento di una soglia, che per noi è altissima, perché dobbiamo superare il 20

Signor Presidente, tre voti di fiducia alla Camera e cinque al Senato: una violenta compressione del Parlamento senza precedenti. Mai un Governo e una maggioranza sono giunti a tanto dal 1861 a oggi, sotto la Repubblica o sotto la monarchia: ben otto voti di fiducia, tra Camera e Senato, sulla legge elettorale, pur di non far votare alcun emendamento.

non dopo cinque ore di discussione, come è avvenuto ieri. Si tratta di un atto di forza che nasconde una debolezza: la paura del voto segreto dei parlamentari della stessa maggioranza. Voi, che avete voluto o deciso questo strappo, continuate a picconare le regole della democrazia parlamentare senza avere la forza o la capacità di costruirne di nuove con il consenso necessario. State creando, in nome della prevalenza del Governo sul Parlamento, dell'urgenza sulla normalità, una costituzione materiale che non trova riscontro nei principi della Costituzione scritta. Procedendo così, contribuite a una crisi della Repubblica senza uno sbocco chiaro, se non una deriva incerta e pericolosa. Un esempio: d'ora in poi una maggioranza qualsiasi potrà cambiare la legge elettorale a pochi mesi del voto, in base alle convenienze del momento e a colpi di fiducia. Per fare cosa poi? Per varare una legge elettorale che non può produrre una maggioranza scelta dagli elettori, che taglia la rappresentanza e che porterà a una pioggia di nominati. Una legge che man mano svelerà i suoi effetti e allargherà il solco tra cittadini e istituzioni. Ci sono i collegi e ci sono le coalizioni, certo. Ma i collegi sono solo un correttivo limitato all'impianto proporzionale e le coalizioni sono coalizioni bugiarde. Sono solo apparentamenti elettorali per avere più eletti, senza l'obbligo di un programma e di un *leader* condivisi. Un *escamotage* che contiene già all'origine il germe della loro dissoluzione. Come ha documentato su «Il Sole 24 Ore» il professor D'Alimonte, questa legge non è in grado di produrre una maggioranza scelta dagli elettori. Sento *leader* politici dire in televisione: dateci il 40 per cento e avremo la maggioranza. È un miraggio. È un sogno. per cento dei seggi nel proporzionale (ed è tanto), per raggiungere i 316 seggi della maggioranza alla Camera una coalizione dovrebbe conquistare ben il 70 per cento dei collegi maggioritari. Un obiettivo impossibile da raggiungere in un sistema multipolare. E poi, le cose non cambierebbero neppure con una percentuale più alta, stratosferica. Con il 45 per cento dei seggi nel proporzionale bisognerebbe conquistare il 65 per cento dei collegi maggioritari. Scenari che hanno le stesse probabilità di realizzarsi di una invasione dei marziani nelle prossime ore. Non è un'opinione, è un semplice calcolo matematico che chiunque può fare. Le coalizioni sono solo uno specchio per le allodole. Il giorno dopo il voto si dovrà andare a un Governo di intese più o meno larghe, probabilmente disarticolando le coalizioni che si sono presentate agli elettori. Questa è la sostanza vera dell'accordo politico che sorregge la legge elettorale.

L'effetto sarà una disillusione di molti elettori e un ulteriore colpo alla credibilità della politica. Se non si voleva o non si poteva andare verso un sistema maggioritario, il Mattarellum, o magari col doppio turno di collegio come in Francia, era meglio allora fare un'operazione verità con gli elettori: scegliere un sistema proporzionale corretto con una soglia del 5 per cento e fare una cosa trasparente. Non è detto che gli esiti per la governabilità sarebbero stati peggiori. Cosi, invece, non avremo una maggioranza e avremo più frammentazione. Ma non finisce qui: l'elezione dei parlamentari si fonda su un sistema a strascico. Se un elettore vota solo il candidato nel collegio uninominale, il suo voto viene assegnato *pro quota* ai partiti della coalizione, anche se non voleva, anche se non si sarebbe mai sognato di votare un partito di quella coalizione. Questa è una grave limitazione della libertà dei cittadini, una violazione dell'articolo 48 della Costituzione. Non a caso, tutti i sistemi elettorali misti hanno il voto disgiunto. In questa legge non è così e solo per rafforzare i partiti che sono in coalizione e il meccanismo dei nominati. Anche il voto bloccato nelle liste dei candidati nella parte proporzionale disegna un legame molto incerto tra elettori ed eletti, perché la scelta degli eletti è in realtà affidata a un meccanismo tortuoso, nazionale e regionale. Altra storia in Spagna, dove si vota su listini corti in circoscrizioni piccole. Ma si dice: non c'erano alternative. Non è vero. Se non Se non si voleva o poteva ritornare a un sistema maggioritario, si poteva ricominciare dal modello tedesco; si poteva lavorare sulle soglie e i premi per armonizzare i sistemi scaturiti dalle sentenze della Corte si poteva perfino lavorare su questo modello, per allargare gli spazi di libertà degli elettori. Invece no: si è perso tempo ed ora il patto non si tocca. Questa non è responsabilità, è solo un calcolo arrogante delle convenienze. elettorale sembra un abito fatto su misura del centrodestra: minimizza le differenze e massimizza i seggi. Meno evidenti le ragioni dell'altro contraente del patto, il PD: il Governo comunque? Il cosiddetto voto utile? Come se le elezioni nazionali e locali non avessero già mostrato che il richiamo al voto utile si è molto indebolito. Vedremo: non sarebbe la prima volta che calcoli presuntuosi si dimostrano sbagliati. sbagliati. Non va bene, comunque, che si faccia una legge elettorale, a pochi mesi del voto, contro qualcuno, contro coloro che non si coalizzano. È un errore grave. Noi di MDP avevamo chiesto almeno di discutere questo disegno la risposta è consistita in cinque voti di fiducia, un macigno deliberatamente messo dal Partito Democratico. Questa legge elettorale segnerà infine un passaggio d'epoca nella politica italiana: viene meno il sogno di una Repubblica che restituisce lo scettro agli elettori. Dopo il Mattarellum, dopo che la Corte costituzionale ha modificato la legge del 2005 e l'Italicum, per ragioni che, inascoltate, erano già state denunciate in quest'Aula, avremo una legge elettorale che in premessa, non come stato di necessità, non può produrre una maggioranza; una legge che sbandiera coalizioni per finta. Avremo elettori che non potranno scegliere direttamente gli eletti. Tutti ingredienti che fanno prevedere un ulteriore scollamento tra cittadini e istituzioni; una responsabilità che lasciamo ad altri, alla maggioranza che nasce oggi e che oggi fa le prove generali per il suo domani. Il no di MDP è un no fermo e convinto. Grazie, Presidente. diversamente dal collega Migliavacca credo che oggi sia un giorno importante per la democrazia italiana e per il nostro Parlamento, perché quest'ultimo farà un passo avanti significativo in quanto consentirà di riaffermare in Italia regole democratiche e di rispettare i principi della partecipazione e della scelta da parte dei cittadini. Evitiamo così lo spettro di una decisione irresponsabile da parte nostra, di una figura pessima quale sarebbe quella di completare la legislatura senza aver dotato il Paese di una legge elettorale che lo metta al riparo da pericolose derive di ingovernabilità. Sarebbero devastanti gli effetti di una mancata approvazione della legge elettorale a pochi mesi dal voto. Una legge elettorale che - lo abbiamo sentito dire da più parti - probabilmente - probabilmente non piace a tutti, non è la migliore, ma ci consente di mettere i cittadini nelle condizioni di scegliere liberamente e senza il rischio di andare al voto con l'attuale sistema assolutamente disomogeneo, incoerente, irrazionale e dunque non applicabile, ancorché rispondente alle decisioni della Corte. Però - lo diceva il collega Quagliariello - la Corte costituzionale si occupa di rettificare le decisioni e le leggi che noi facciamo in Parlamento, non si occupa certamente di scrivere le leggi. Quindi uno strumento di democrazia così importante come la legge elettorale non può che essere scritto dal Parlamento, l'unica sede attraverso la quale gli elettori decidono la propria rappresentanza. quindi sottrarci a quello che deve essere un vero e proprio dovere per tutti noi e non una semplice scelta. È una legge scritta con l'accordo dei partiti che rappresentano, in parte, la maggioranza e, in parte, l'opposizione; un accordo necessario, ma non per questo generato da forzature, La tecnica è nota: quella di dire sempre «no», per creare artificiosi motivi, utili a rendere calda la campagna elettorale o trovare argomentazioni che possano animare le piazze. spesso in maniera troppo sbrigativa, viene tacciata di incostituzionalità, un termine forte che fa presa sulla gente e sui cittadini che devono valutare, ma che non ha fondamento alcuno, perché tutti tutti gli esperti e i costituzionalisti che abbiamo ascoltato nelle varie Commissioni si sono espressi in maniera critica, con osservazioni e e con riferimenti al dettato costituzionale, ma senza fare rilievi evidenti di incostituzionalità. Si può dire che è una legge che a qualcuno piace e ad altri meno, ma sulla coerenza costituzionale non ci sono dubbi. È una legge che comunque è venuta fuori da un dialogo, da una mediazione tra le diverse esigenze della maggioranza dei Gruppi politici e parlamentari che rappresentano il popolo in Parlamento. Questo è il metodo per scrivere le regole: lavorare insieme per contemplare una serie di princìpi espressi dalle varie parti politiche in un contesto di coerenza normativa e compatibilità costituzionale. Una legge che garantisce rappresentatività, governabilità, possibilità di scelta da parte degli elettori. Il bilanciamento tra quota proporzionale e maggioritaria, rispettivamente di due terzi e un terzo, garantisce agli elettori, attraverso la previsione dei collegi uninominali sia alla Camera che al Senato, di scegliere il proprio candidato e il proprio deputato di collegio. Il rapporto tra il parlamentare e il territorio credo che sia indispensabile, un elemento fondativo della rappresentatività. Si è molto discusso sulle preferenze e sulle liste bloccate e questi saranno motivi di attacco

perché ne conosciamo gli effetti distorsivi, soprattutto noi parlamentari - lasciatemelo dire - del Meridione. Se vogliamo che il sistema delle liste bloccate più corte, quindi con i candidati più riconoscibili rispetto al Porcellum, non appaia un esproprio nella facoltà di scelta nell'espressione del voto, è necessario che i partiti si organizzino per metodi di scelta e di selezione dei candidati più partecipati e trasparenti ed è in discussione un disegno di legge, di cui sono relatore insieme al collega Mirabelli, che mi auguro possa vedere la luce al più presto. Il problema si trasferisce quindi alla volontà dei partiti, che hanno la responsabilità delle scelte, così come avviene, d'altronde, in Germania. Sono state introdotte le coalizioni, quelle che l'Italicum aveva cancellato con il premio alla lista. Una delle critiche più feroci che si rivolgevano a quella legge era quella del pericolo dell'uomo solo al comando. Noi siamo sempre stati sostenitori di un sistema di aggregazione in coalizione sotto un programma comune. Poi, il giudizio sulla validità del programma e sulla coerenza delle coalizioni lo daranno i cittadini, gli elettori e non i censori, che usano questi argomenti per alimentare proteste inutili e strumentali. Il sistema delle coalizioni e delle aggregazioni di questo tipo, quindi, non può non essere riconosciuto come virtuoso. la coerenza dei partiti su programmi chiari e condivisi, con piattaforme programmatiche solide e di respiro valoriale, non è convincente, si alimenta la convinzione che la possibilità di un futuro Governo di larghe intese sia un disegno preventivo, un cosiddetto inciucio, e non una una delle opzioni di Governo in caso di stallo politico delle Camere. Signor Presidente, ci apprestiamo a dotare finalmente il nostro Paese di una legge elettorale fondata su regole certe; regole che servono all'Italia per dare concretezza alle istituzioni e garanzia agli osservatori esterni, che ritengono prevalente il rischio della ingovernabilità, della tenuta politica, rispetto spesso a quello economico e finanziario. Ciò non ci ha portati a scrivere una legge elettorale qualunque essa sia, ma una legge che ha elementi fondanti coerenti con il con il desidero di restituire credibilità e dignità alla politica e migliorare il rapporto tra gli italiani e le istituzioni. Per questo motivo, signor Presidente, il Gruppo di Alternativa Popolare, che ha avuto un ruolo attivo e propositivo nella costruzione di questa legge, voterà

cari colleghi, sono passati sessantaquattro anni dall'unica volta in cui il Senato ha dovuto subire l'umiliazione del voto di fiducia su una legge elettorale. Ma quella legge fu approvata con la fiducia solo al Senato; non era mai accaduto, prima di oggi, che una legge elettorale fosse imposta a colpi di fiducia in entrambi i rami del Parlamento. sessantaquattro anni, la legge approvata all'inizio del 1953 ha sempre mantenuto il titolo poco onorifico di «legge truffa», ma oggi è destinata a perdere lo scettro. Questa legge, infatti, è tanto disonesta e truffaldina che andrebbe chiamata non Rosatellum-*bis* ma Truffarellum-*bis.* Pensavamo che dopo il risultato straordinario del *referendum* del 4 dicembre ci fosse una riflessione, che la lezione fosse servita. Pensavamo, in tutta onestà e in buona fede, che questo avrebbe spinto a costruire un modello di legge elettorale pienamente costituzionale, cioè ispirata pienamente ai principi costituzionali. Invece, con questa legge, voi ingannate scientemente e freddamente gli elettori, chiedendo loro di votare per coalizioni che sono puri ologrammi, destinate a dissolversi un attimo dopo aver rubato i voti. Le coalizioni disegnate da questa legge ricordano quei matrimoni di convenienza nei quali i coniugi si presentano con in tasca già pronte le carte per il divorzio; subito dopo la cerimonia si spartiranno i regali e chi si è visto si è visto. Alla faccia degli elettori, beffati per l'ennesima volta. Ma forse era proprio quello che si voleva. Dopo cinque anni spesi a parlare a vanvera, da parte di alcuni, del diritto degli elettori a scegliere i loro rappresentanti, sta per essere servita a quegli elettori una legge in cui, alla fine, forse neanche un parlamentare verrà scelto liberamente e direttamente dai cittadini. Le Camere saranno occupate per intero dai nominati, cioè dai fedelissimi delle varie segreterie. segreterie. Dopo decenni passati a parlare del necessario e urgentissimo riequilibrio della rappresentanza di genere, viene ammannita una legge che, alla fine, per ogni donna eletta, porterà in Parlamento quattro maschi. In compenso, però, viene introdotta una novità che nessuno, devo dire, nel 1953 avrebbe osato prendere in considerazione: grazie all'espediente di negare la possibilità del voto disgiunto, o meglio attraverso il voto unico per due diversi sistemi elettorali, maggioritario e proporzionale, alcuni voti, voti sono del genere supermercato: paghi uno e prendi tre.

Si violano così, in un colpo solo, i principi del voto eguale, libero, personale e diretto sancito dalla nostra Costituzione (articoli 3, 49 e 56).

impone, su mandato di un segretario di partito prepotente e arrogante, non è solo una truffa: è un monumento all'irresponsabilità. Tutti sapete che è una legge fortemente esposta al rischio di incostituzionalità. Tutti sapete che la terza bocciatura consecutiva di una legge elettorale da parte della Corte costituzionale implicherebbe il discredito definitivo delle istituzioni democratiche, ma non vi importa, perché tanto a quel punto le elezioni ci saranno già state. Del resto, come ha segnalato persino il senatore Giorgio Napolitano ieri nel suo intervento, anche senza la bocciatura della Corte costituzionale questa legge dovrà comunque essere cambiata di nuovo. L'eventualità che all'indomani delle elezioni non sia possibile dar vita a nessuna maggioranza di Governo è del tutto realistica e, anche se per miracolo così non sarà, si tratterà comunque di una maggioranza spuria, fragile, oppure forse era proprio questa l'intenzione: arrivare con questa legge elettorale alle larghe o strette intese. Per anni ci avete ossessionato con discorsi secondo cui si poteva anzi, si doveva sacrificare una parte della rappresentanza in nome della governabilità e infatti con questa legge è stata sacrificata, sì, la rappresentanza, ma senza neppure ottenere risultati sul fronte della governabilità: un capolavoro!

un Parlamento chiamato solo a ratificare decreti a colpi di fiducia e alla fine con un unico obiettivo: l'abbattimento dei diritti, tanto quelli dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente, quanto quelli del Parlamento. In questa legislatura si è reso istituzionale e permanente il precariato, sono stati smantellati i diritti dei lavoratori, a partire dalla cancellazione dell'articolo 18. Sono stati difesi gli interessi della finanza e delle banche a scapito di quelli dei cittadini e dei risparmiatori. Avete approvato lo sblocca Italia, umiliato la scuola pubblica con la buona scuola, si sono fatte passare le organizzazioni non governative, impegnate a salvare vite, per criminali (vedo qui Minniti) e potrei continuare con un lungo elenco, tentando di costringere sempre al silenzio tanto i cittadini quanto il Parlamento, al quale ormai lasciate solo il compito di «obbedir tacendo». Il voto del 4 dicembre scorso dovrebbe aver dimostrato che non è possibile imbavagliare un popolo e ignorarne la volontà troppo a lungo. A Renzi e Berlusconi, i due capi partito che con questo inganno sperano di evitare un tramonto che sentono incombere, voglio ricordare che il solo esito della legge imposta con la fiducia 64 anni fa fu il declino del *leader* che l'aveva voluta, De Gasperi (e mi scuso per il paragone ardito). L'imbroglio ai danni degli elettori che state perpetrando non vi porterà fortuna.

È in balia di un vero proprio scollamento dalla realtà che si era già palesato con il *referendum* del quattro dicembre scorso, che era convinto di vincere a mani basse. Non vede quel che succede in Italia, non vede un disagio sociale che cresce, nonostante le favole rassicuranti su una ripresa di cui nessuno si accorge. Non vede quel che succede alla nostra democrazia, vicina ad essere sommersa dal discredito e dalla sfiducia. Non vede quel che succede in Europa, dove monta sempre di più un'ondata minacciosa, provocata in buona parte proprio da politiche di questo genere, dal fatto che i cittadini sentono di non contare più nulla e si dibattono nelle spire di una crisi che è finita solo sulla carta. *(Brusio)*. il brusìo è continuo (per quanto io sia abbastanza allenata). Di fronte a questa deriva e a questa situazione drammatica, credo che noi, Sinistra, abbiamo il dovere non solo politico ma anche etico e morale di mettere in campo un'alternativa reale, radicale

che minaccia di trascinarlo a fondo. Fatevela la vostra coalizione con i Verdini e con gli Alfano e con qualche altra lista civetta, ma questo non vi salverà, questa volta il ricatto del voto utile non funzionerà. Solo la presenza di un quarto polo e di una Sinistra unita, plurale e radicalmente alternativa al PD e alle sue politiche scellerate di questi anni può ridare voce e speranza ai giovani, alle donne, ai lavoratori e ai precari che hanno pagato e continuano a pagare sulla propria pelle il prezzo di queste politiche. I senatori di Sinistra Italiana, Presidente, colleghi, voteranno no, fortemente no a questa legge truffa e su di voi, Partito Democratico, ricadrà ancora una volta, come avete fatto cercando di scassare la Costituzione, l'onta di questo ennesimo schiaffo alle regole democratiche e alla nostra Costituzione.

la luce della democrazia resa più fioca. È su questa penombra che contano i ladri, che adesso cercano di staccare definitivamente i fili, disattivare i sistemi di sicurezza e impadronirsi del voto dei cittadini. E punto il dito sul Partito Democratico, con la gongolante complicità di Forza Italia e Lega! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non i loro elettori, ma questa nomenclatura di nominati, tronfi della loro maggioranza fasulla, gonfiata da una legge incostituzionale, il Porcellum. E questa arroganza l'abbiamo vista all'opera. Cose mai accadute, almeno in epoca repubblicana. Sono almeno cinque i piccoli, grandi *golpe* - vedeteli come vi pare, a seconda della convenienza - del partito unico: il primo, in apertura di legislatura, la rielezione inusitata a Presidente della Repubblica di Giorgio Napolitano, il pilota automatico che ha garantito il vostro sistema di potere, mentre fuori dal palazzo i cittadini, anche della vostra parte, invocavano il nome di Rodotà. Il secondo, nel 2015, l'imposizione di un'altra legge elettorale a colpi di fiducia, l'Italicum, anch'essa incostituzionale. Siete recidivi. È il vostro marchio di fabbrica. L'avete concepito ad arte solo per una Camera, generando il *caos*: voi siete pericolosi! Il terzo: stravolgere la Costituzione a colpi di mano, tagliole, rimozione di senatori dalla Commissione. Vi siete risvegliati il 4 dicembre, seppelliti dai 20 milioni di voti di chi ha preferito la Costituzione di Pertini e Calamandrei a quella di Renzi, Boschi, Verdini e Alfano. Il quarto: avete razzolato voti ovunque, tra oltre 500 voltagabbana e Gruppi parlamentari escogitati *ad hoc*, con la parte più becera del centrodestra. Con loro avete condiviso tutte le leggi vergogna, coperte con nomi ingannevoli: il *jobs act*, che ha condannato i giovani al precariato o a emigrare; la buona scuola, che ha messo sotto ricatto i professori italiani; lo sblocca Italia, che ha regalato i nostri mari ai petrolieri; la Boccadutri,

Il quinto *golpe* è in atto: quello che voi avete chiamato Rosatellum, per occultare la paternità di Verdini, trucca di nuovo le regole del voto, a pochi mesi dalle elezioni, per consentire a un gruppo di capibastone di nominarsi i due terzi delle prossime Camere, con otto voti di fiducia!

"compagni" del PD, vi riconoscete ancora tali? Con due fiducie su due leggi elettorali diverse, avete doppiato Mussolini. Dovreste essere incriminati per apologia del fascismo! Ma qui non c'è nemmeno ideologia: questa legge sottende un'idea della politica meramente affaristica e consociativa. Viene da quella parte del PD, allora Democratici di sinistra (DS), che nel 2003 rivendicava, candidamente, di avere garantito a Berlusconi di non toccare il suo conflitto di interessi. È il PD che, all'inizio di questa legislatura, ha architettato, con malcelato entusiasmo, il Governo insieme a Berlusconi, che in questi anni, per collusione o ignavia, ha aperto furtivamente le porte alle leggi vergogna, ai compromessi sulla giustizia, quando non addirittura disattivando o insabbiando le leggi antimafia e anticorruzione, che si è apparentato in tre Governi con emissari berlusconiani, come Alfano, Lorenzin, Lupi e Cicchitto. È lo stesso partito che oggi regala a Berlusconi - che è ancora qui, come convitato di pietra la migliore legge elettorale possibile per lui, che produce il *caos* per un intero Paese, mentre lui, servito da una truppa fedele di nominati, avrà miglior agio di agire nel torbido. In un sol colpo avete reinsediato un pluricondannato in via definitiva a capo di una forza politica. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Gli consentite ancora la vergogna delle liste bloccate, avete progettato ammucchiate elettorali per puro interesse e previsto l'ingovernabilità più totale, per giustificare il vostro tentativo di ricostituire il partito unico renzusconiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per ottenere questa apoteosi dell'orrore, avete piegato l'elettore: il voto apposto salta, a tradimento, da un nome a una lista, da una lista a un nome, da una lista a un'altra lista, da un collegio uninominale a uno plurinominale, da un collegio del Nord a uno del Sud e viceversa, come una pallina da *flipper*, ma peggio, come una *slot machine*: tu pigi il bottone e credi di scegliere, ma c'è un *software* che decide al posto tuo e ti mangia i soldi. *(Commenti dal Usate questo schifo per allontanare i cittadini dal voto, su questo conta Berlusconi. Ma quale Rosatellum? Questa è la legge «bunga bunga»: un'orgia di pluricandidati, dove tutti vanno con tutti! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. In cui l'utilizzatore finale è drammaticamente sempre lo stesso. Ma non vi vedete? Siete due bande, la stessa banda, la medesima concezione di un Paese suddito. *(Commenti dal Gruppo PD).* Voi, senza idee, senza programmi, ma con il medesimo progetto: mantenere le poltrone e il potere a vostro uso e consumo, per continuare a spolpare e a sfinire una Nazione allo stremo. Avete compiuto con questa legge l'orrenda mutazione che ha trasformato destra e sinistra nelle due facce della stessa banconota. Lo vedranno tutti alla votazione finale: le luci "verdine" che si accenderanno a breve sui *display* mostrano il senso di questo incrocio di interessi inconfessabili, in cui - ascoltate bene la Lega di Salvini voterà allo stesso modo di Alfano e di Verdini, Gasparri voterà come Zanda, Scilipoti voterà come la Finocchiaro, questa voterà come Casini e Casini come Calderoli! La Lega, che chiede maggiore autonomia nelle Regioni, sta contrattando il ritorno all'ovile con Berlusconi, che l'autonomia gliel'ha già bocciata nel 2008. *(Applausi che si riempie la bocca di tutela delle minoranze, in Alto Adige aveva già pronta la legge truffa per fare diventare l'SVP il pigliatutto e prevaricare le minoranze nella sua Provincia! *(Applausi dal Il nostro no a una vergognosa riscrittura delle regole elettorali è quindi un dovere politico e morale. Presidente, davanti alle macerie che stanno lasciando all'Italia, il Movimento 5 Stelle assume su se stesso una missione. Una missione non di forza o di arroganza, ma di progresso, di civiltà e di verità. Il Movimento 5 Stelle presenta il primo programma di Governo costruito direttamente dai cittadini per i cittadini, che riporterà l'Italia a essere un Paese normale. La partitocrazia (PD, Forza Italia, Lega, Alfano) si sta apparecchiando la tavola per la grande abbuffata: ma davvero pensate di combattere le idee con le poltrone? Non si ferma chi non si arrende mai! Sbarrando il corso di un fiume non fate che alzarne il livello; la democrazia liquida arriva al mare. L'ultimo pensiero è per i cittadini italiani che ci guardano da fuori: dipende da voi, soltanto da voi. Aprite gli occhi, informatevi, state attenti. E alle prossime elezioni si ripeterà quello che abbiamo già visto il 4 dicembre 2016: ci dipingevano pochi e rassegnati, siamo stati 20 milioni e abbiamo stravinto. Ora, nel giorno più buio della democrazia, alziamo insieme lo sguardo e guardiamo oltre. Italia, tornerai libera, tornerai grande!

Forza Italia ha tenuto in tutto il percorso parlamentare di questo disegno di legge elettorale una posizione chiara e trasparente. Abbiamo partecipato attivamente alla stesura del testo e lo sosteniamo convintamente in questo ultimo voto. Un sostegno che, ovviamente, si limita al sistema elettorale, ed è per questo che ieri non abbiamo preso parte ai voti di fiducia sugli articoli, non volendo e non potendo dare la fiducia a questo Governo. Un Governo del quale non condividiamo le politiche economiche, fiscali e del lavoro; un Governo che, nonostante alcune iniziative, che rimangono e sono rimaste isolate ed estemporanee, riteniamo debole in politica estera e in Europa. Un Governo espressione chiaramente della sinistra di questo Emiciclo, al quale come centrodestra ci sentiamo e siamo alternativa. Saranno finalmente i cittadini a scegliere, nella ormai prossima scadenza elettorale, il Governo del Paese,

- al contempo - a garantire stabilità al prossimo Governo, pur in assenza di un premio di maggioranza che, nell'attuale quadro politico, rischierebbe di alterare fortemente il voto. Questo sistema è in grado di determinare una semplificazione dell'offerta politica. In un quadro tripolare, dove una coalizione sperimentata e a vocazione governativa come il centrodestra si confronta con la sinistra, divisa oggi tra maggioranza e opposizione, e con un partito che ha fatto della protesta l'unica proposta, è responsabilità del Parlamento e di quest'Assemblea consentire ai cittadini di esprimersi attraverso un voto che sia poi rispettato con la formazione di un Governo stabile. La presenza di ragionevoli soglie di sbarramento e la naturale agevolazione al formarsi di coalizioni contrastano in maniera efficace l'endemica abitudine alla frammentazione del sistema politico italiano; un fenomeno che non sempre siamo riusciti a evitare, nemmeno all'interno del quadro tendenzialmente bipolare che ha caratterizzato gran parte della cosiddetta seconda Repubblica, pur potendo vantare una durata dei Governi nettamente superiore, in media, a quelli della prima Repubblica. Questo sistema non regala voti per blindare maggioranze di Governo (e sarebbe improprio in uno scenario così diviso), ma descrive in maniera fedele le scelte dell'elettore

dato a chi ha ottenuto semplicemente una manciata di voti in più degli altri, ma un riconoscimento alla proposta politica che più convince il cittadino, con donne e uomini competenti e stimati, capaci di amministrare e governare. Mi verrebbe da dire un disegno di legge giusto, equilibrato e rispettoso che, grazie al meccanismo uninominale, premia chi è conosciuto, stimato e apprezzato sul territorio. Il voto di oggi rappresenta un atto di responsabilità che vede forze politiche della maggioranza e dell'opposizione approvare insieme un disegno di legge elettorale che trova la contrarietà solo di chi non confida nella propria credibilità di fronte agli elettori. Non abbiamo timori nel condividere questo voto anche con la maggioranza di Governo. Non li abbiamo perché ogni critica che può essere legittimamente mossa contro il testo in esame non può metterne in discussione la costituzionalità.

Non li abbiamo perché abbiamo un'identità politica chiara, definita e riconosciuta dai nostri elettori. Non li abbiamo soprattutto perché conosciamo il valore delle istituzioni sappiamo bene che il nostro compito, quello che ci hanno assegnato i cittadini, è onorarle lavorando nelle Commissioni e nelle Assemblee parlamentari e non umiliarle con comportamenti inadeguati a questi luoghi, nel totale spregio di quei cittadini che in quest'Aula

Non li abbiamo, infine, perché riteniamo un giusto proposito ridare la parola agli italiani, rispettare la volontà dell'elettore e consentire allo schieramento scelto attraverso il voto di vincere e governare. Noi vogliamo vincere e governare e siamo convinti che la nostra proposta, quella di un centrodestra ampio e coeso, sia la migliore per l'Italia. Valorizzeremo i nostri uomini e le nostre donne che, grazie al lavoro in Parlamento, sul territorio e nelle amministrazioni locali, hanno acquisito il merito e la possibilità di consegnare alla propria passione politica un impegno costituzionale ancora più alto.

per interessi di partito e tensioni che esulavano dal tema in discussione. Forza Italia, però, ha dimostrato in ogni passaggio la capacità e la fermezza di forza responsabile e pragmatica, volta in ogni momento ad agevolare l'accordo del maggior numero possibile di soggetti per scongiurare il pericolo di andare al voto con il frutto delle sentenze della Consulta, condannando il Paese all'instabilità, emendando due leggi già in partenza incompatibili fra di loro. Ricordo, infatti, che il cosiddetto Consultellum del Senato era ciò che restava del Porcellum, mentre per la Camera la sentenza interveniva sull'Italicum. La Corte quindi, senza alcuna volontà legislativa, lasciava suo malgrado due sistemi completamente contrapposti: alla Camera, un premio di maggioranza, capilista bloccati e soglia di sbarramento bassa, al 3 al Senato, preferenze, coalizioni e sbarramenti alti. Siamo convinti che la legge che stiamo per approvare sia il miglior risultato possibile allo stato attuale, ma non avremmo avuto timore a confrontarci con un altro sistema, se fosse stato l'unico su cui far convergere una maggioranza più ampia di quella del Governo. Le leggi elettorali, signor Presidente, si sono sempre scritte insieme. Non abbiamo mai anteposto i nostri interessi di parte all'obiettivo primario: dare al Paese una legge che fosse omogenea fra Camera e Senato, che rispettasse le sentenze della Corte costituzionale, ma che fosse frutto del potere legislativo del Parlamento, il luogo in cui i cittadini sono rappresentati. Questi sono i principi e i valori su cui si basa una Repubblica parlamentare e oggi in quest'Aula scriviamo, per conto dei nostri cittadini, una buona pagina della storia della nostra Repubblica. Stiamo ponendo le basi perché la prossima sia una legislatura fedele alla volontà degli italiani, espressa con il voto, rispettosa delle regole della democrazia e capace di dare al Paese vigore e prospettive. La protesta, signor Presidente, sta nel passato; la proposta sta nel futuro. Dimostriamo di essere capaci di rispettare le regole con cui i nostri padri fondatori hanno scritto per noi un passato glorioso, per scrivere tutti insieme il nostro futuro.

voglio iniziare ricordando che in materia di legge elettorale ci sono due punti sui quali l'Assemblea del Senato dovrebbe raccogliere l'unanimità. Il primo è che quella elettorale è una legge fondamentale della democrazia e il secondo è che per più di vent'anni l'Italia non è stata capace di darsi una buona legge elettorale. Non sto parlando di una legge elettorale perfetta, che non esiste, né di una legge in grado di accontentare tutti, ma almeno di una stessa legge per Camera e Senato, votata da maggioranza e opposizione. Se partiamo da qua, diventa chiaro che il senso del voto che stiamo per esprimere va ben oltre l'interesse dei nostri partiti e riguarda invece il funzionamento della democrazia e del Parlamento, che non può permettere la casualità

Sul finire del 2013 il deputato democratico Giachetti arrivò persino allo sciopero della fame per sostenere il ritorno al Mattarellum. Il tentativo andò a vuoto per l'opposizione di molti, anche del mio partito, persino di tanti che oggi, fuori tempo massimo, chiedono che si ritorni proprio a quel Mattarellum che allora non aiutarono a portare in Lo stesso copione si è ripetuto pochi mesi fa, quando ripetutamente il Partito democratico ha riproposto il Mattarellum nell'indifferenza generale, con l'eccezione della posizione di un nostro avversario politico, la Lega Nord. Come pure ancora bruciano gli applausi nell'Aula della Camera per la bocciatura a scrutinio segreto di un importante emendamento al proporzionale alla tedesca. La maggioranza era molto larga, ma i franchi tiratori hanno vinto lo stesso. Oggi, anche chi ha cantato vittoria per quell'emendamento bocciato chiede di tornare al proporzionale di cui ha festeggiato la fine. Queste vicende parlamentari non aiutano, onorevoli senatori, ma ora siamo al momento della verità, alla fine della legislatura, e tra poco il nostro voto dividerà l'Assemblea non tra destra e sinistra, non tra maggioritari e proporzionalisti, ma tra chi vuole che si vada a votare non con una legge del Parlamento, ma con gli effetti di due sentenze della Corte costituzionale e chi, al contrario, vuole un'unica legge in modo che le due Camere abbiano una composizione omogenea. Conoscete bene il contenuto della legge che prende il nome dall'onorevole favorisce la rappresentanza dei territori e la formazione di quelle coalizioni che servono ai partiti per rafforzare i legami politici. Con i collegi uninominali e quelle liste di soli quattro candidati, che la Corte ha suggerito per renderli identificabili, la legge tiene insieme le caratteristiche del proporzionale e del maggioritario. La legge è il frutto di un delicato lavoro di mediazione tra forze di maggioranza e di opposizione, forze molto diverse e con interessi diversi. In Parlamento, quando si fanno proposte di modifica, sarebbe bene che chi le avanza spieghi bene da quale nuova maggioranza verrebbero approvate perché, diversamente, è solo ordinaria propaganda. *(Applausi

non dal 2013, come ho ascoltato, ma dal 2011, con il Governo presieduto dal professor Monti, la frantumazione parlamentare non consente maggioranze omogenee né di destra né di sinistra. Da allora, per questa ragione, abbiamo avuto Governi sostenuti da partiti dei due schieramenti. È sorprendente che molti che oggi strillano siano stati tra i promotori di quelle alleanze e abbiano sostenuto quei Governi. *(Applausi dal L'Italia ha assoluto bisogno che la legge di bilancio venga approvata. Se non lo fosse, andremmo all'esercizio provvisorio e non voglio nemmeno pensare quali sarebbero le conseguenze per i lavoratori, per le famiglie e tutti i cittadini. È mia opinione che le forze politiche che concorreranno all'approvazione della legge bilancio mostreranno di fronte al Paese con questo atto senso di responsabilità. Il dibattito che ha accompagnato la gestazione della legge Rosato rappresenta un esempio di come una cattiva discussione può impedire qualsiasi intesa. Abbiamo sentito dire che il presidente Gentiloni è peggio di Mussolini e che i parlamentari che stanno approvando la legge altro non sono che un manipolo di eletti. Ho sentito diversi senatori parlare di Fascistellum. Siamo abituati ad una polemica politica fatta di volgarità e di insulti gratuiti, ma dobbiamo darci un limite. Due giorni fa abbiamo visto in quest'Aula una pianificata occupazione dei banchi del Governo, che sono certo verrà debitamente sanzionata. La violenza fisica in Aula è l'opposto della democrazia. Spintonare e strattonare i collaboratori parlamentari, che ringrazio molto per il loro difficile lavoro

Un Parlamento che accetti, senza reagire e difendersi, che al suo interno l'attività legislativa venga interrotta e minacciata con la violenza è un Parlamento che deve seriamente interrogarsi sul suo funzionamento. Le frasi sul fascismo e Mussolini, più che un insulto al presidente Gentiloni Silveri, umiliano chi il fascismo lo ha conosciuto davvero e tutti i veri antifascisti che sanno ben valutare le differenze tra allora e oggi. Lo dico molto seriamente ai parlamentari dell'opposizione che usano questo linguaggio. Ma come intendete il dibattito politico in Parlamento? Se evocate con tanta leggerezza il fascismo, vuol dire che non avete capito quale tragedia il fascismo è stato per l'Italia. Pensate veramente che ci sia una briciola di valore politico positivo nel discutere in questo modo di legge elettorale? E chiedo: come vedete il futuro politico del nostro Paese? Come vedete il vostro stesso futuro se lo anticipate paragonando Gentiloni Silveri a Mussolini? Siamo abituati a sentir dire che le leggi elettorali sono le più politiche tra tutte le leggi. È un'espressione che può essere intesa in vari modi, ma quando il consenso o l'opposizione alla legge riflettono l'idea che quella legge ci aiuterà a vincere o la paura che sarà lei a farci perdere le elezioni, allora si tratta di cattiva politica. A chi voterà contro la legge perché teme la sconfitta elettorale e a chi voterà a favore pensando di avere già vinto, dico di non fidarsi né dei sondaggi, né delle simulazioni e nemmeno delle fantasiose previsioni del senatore Calderoli. Il vero sondaggio lo faremo i primi mesi del 2018,

Candiani)*. Nessuna legge elettorale è riuscita a far vincere chi non ha i voti o a far perdere chi i voti li ha. Con il famigerato Porcellum, pensato apposta nel 2005

ha una composizione molto diversa da quella che avevano annunciato i sondaggi. Lo sa bene il Movimento 5 Stelle, di cui nel 2013 nessuno aveva previsto i tanti consensi che ha ricevuto e che poi ha sprecato con un'attività parlamentare inutilmente rumorosa e persino violenta. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Eletti tutti con un *click*, hanno perso metà dei senatori e ancora di più ne perderanno alle prossime elezioni. Lo ripeto: il vero sondaggio lo faremo con il voto all'inizio del 2018. Negli ultimi giorni, però, una questione ha tenuto il campo e non voglio eluderla: se sia corretto approvare una legge elettorale con i voti di fiducia. Tralascio ogni osservazione su come negli ultimi decenni tutti i Governi abbiano sentito la necessità di usare con fermezza il voto di fiducia nel tentativo di porre rimedio alle difficoltà della capacità decisionale del Parlamento. Ne ha fatto cenno ieri il presidente Napolitano, e io debbo ricordare che si sono trovati in questa necessità i presidenti Berlusconi, Prodi, Monti, Letta, Renzi e, da ultimo, Gentiloni. Tutti, proprio tutti, i Presidenti degli ultimi venticinque anni. Lo dico a malincuore, ma con il nostro bicameralismo paritario e con un sistema politico così frammentato, la fiducia è diventata di fatto uno strumento abituale, usato da tutti i Governi di destra o di sinistra, nel tentativo di far funzionare, come possibile, istituzioni molto traballanti. Per queste ragioni i Governi degli ultimi anni hanno posto la fiducia non solo su provvedimenti di propria iniziativa, ma anche su disegni di legge parlamentari. In questa legislatura è stata approvata con fiducia la legge sulle unioni civili, che pure era di origine parlamentare. E non appena avremo la certezza di avere i voti necessari, accoglierei con molto favore una decisione del Governo di mettere la fiducia sullo *ius soli*, che non èun provvedimento del Governo, prima della fine di questa legislatura. È stato detto però che non si approvano con fiducia le leggi elettorali. 35 di quest'anno la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i rilievi sollevati sulla decisione di porre la fiducia su leggi elettorali. Dunque, se siamo dentro la Costituzione, chiedere o non chiedere la fiducia è un atto squisitamente politico e così lo dobbiamo giudicare. Dobbiamo valutarlo anche tenendo conto della delicatezza e dei rischi connessi all'attuale momento istituzionale, ordinamentale e politico. di non sapere che l'Italia solo ora sta uscendo da una crisi economica e sociale che dura da più di dieci anni e che per non tornare indietro ha bisogno di un Parlamento almeno omogeneo nella composizione delle due Camere? Possiamo correre il rischio che uno sgambetto, con il voto segreto, ci faccia andare al voto con due leggi profondamente diverse? Possiamo indebolire ulteriormente il nostro Parlamento in una fase internazionale nella quale i rischi della pace sono altissimi e si è persino riaffacciata la minaccia atomica? Possiamo andare in Europa, cercando di far valere i nostri diritti, con un Parlamento eletto con due leggi diverse? Se debbo dirvi la mia opinione, con più di cento voti segreti, costruiti, come si è visto, per favorire gli agguati, il voto di fiducia alla Camera dei deputati ha avuto molto semplicemente il valore di far votare a scrutinio palese una legge importante che, al contrario, come già è accaduto, sarebbe certamente caduta in una delle trappole dei voti segreti. *(Commenti dai Gruppi che per come si è ridotto il voto segreto io sono fermamente contrario al suo uso. Non è più voto di coscienza, ma è un voto di manovra politica. *(Applausi Lo dimostra il fatto che siede qua un movimento che si è sempre dichiarato contro il voto segreto e per favorire gli agguati su questa legge anche ieri ha chiesto il voto segreto. Al Senato la fiducia è stata non solo una decisione egualmente necessaria, ma anche un'assunzione di responsabilità politica, non solo perché, veramente irresponsabilmente, sono stati presentati al Senato una cinquantina di emendamenti suscettibili di voto segreto e visibilmente strumentali, ma anche per la necessità di non sovrapporre la legge elettorale alla legge di bilancio. Le senatrice e i senatori del PD voteranno la nuova legge elettorale e lo faranno in considerazione del suo contenuto, ma anche ben sapendo che oggi tra noi la divisione è tra chi lavora per dare stabilità a una nuova legislatura, composta da due Camere in modo omogeneo, e chi lavora pensando di poter trarre qualche vantaggio politico da due diverse leggi elettorali, mai approvate dal Parlamento e destinate a produrre impotenza parlamentare e debolezza di Governo. *(Applausi

è chiaro che ci troviamo di fronte a un Governo che, insieme ai suoi alleati parlamentari, marginalizza i quasi cinque milioni di cittadini italiani residenti all'estero, da oggi, cari colleghi, cittadini di serie B. Dopo aver degradato la rete consolare, oggi assistiamo al tentativo di colpire anche la credibilità del voto all'estero. Questo Governo ha infatti deciso di dare agli italiani residenti in Italia la possibilità di candidarsi anche all'estero, negando invece ai cittadini del collegio estero la possibilità di candidarsi in qualsiasi

Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge il divieto di potersi candidare all'estero per tutti coloro che abbiano ricoperto una carica di Governo (ellettiva o no) nel Paese di residenza nei cinque anni precedenti. Ancora una volta, signor Presidente, cittadini di serie B. Magari, signor Presidente, qualche futuro candidato nel più grande Paese sudamericano si sente minacciato politicamente per via di questa manovrina?

a una legge elettorale che sembra corrispondere più a contingenti esigenze politiche che a un sostenibile disegno istituzionale. Questa legge, infatti, non soddisfa nessuna delle due finalità proprie di un modello elettorale (la rappresentanza e la governabilità), né realizza un ragionevole equilibrio tra loro. La rappresentanza è criterio prevalente nel nostro dettato costituzionale e condurrebbe molti elettori a ritornare al voto con lo scopo di scegliere il proprio partito, i propri principi, la propria cultura politica, i propri parlamentari, meglio ancora se con voto di preferenza, a votare insomma per e non contro un progetto politico. È invece facile supporre che la correzione maggioritaria disincentivi questa propensione, inducendo larghe coalizioni, senza peraltro premiarle al punto da risultare autosufficienti per il futuro Governo. In questo modo si produce la situazione assurda per cui la legge contemporaneamente incoraggia una coalizione e ne programma la dissoluzione il giorno successivo al risultato, pena il ritorno immediato alle urne, con l'effetto di rendere colpevole di fronte agli elettori e fragile nei contenuti di Governo un eventuale compromesso tra forze politiche che si sono contrapposte nella campagna elettorale. D'altronde, perché dovrebbe funzionare domani quell'incontro fra sinistra e popolari che non ha funzionato in questa legislatura? Divisivi sono stati infatti tutti i provvedimenti che non hanno assorbito ma esaltato la nostra più che ventennale anomalia giudiziaria; divisive sono state le leggi eticamente sensibili, cui spero non se ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane; insoddisfacenti sono risultati gli stessi provvedimenti economici e sociali, perché non hanno ridotto il nostro ritardo rispetto agli altri maggiori Paesi dell'Unione. Temo quindi di essere facile profeta ipotizzando presto una nuova legge elettorale, ma i costi in termini di fiducia nella nostra democrazia potrebbero essere nel frattempo molto elevati.

per giunta a pochissimi mesi dalle elezioni; una legge elettorale frutto dell'ennesimo inciucio dietro le quinte e che perpetua una classe politica che alimenta questo sistema disastroso. I soliti partiti faranno il lavoro sporco dell'Unione europea, facendo credere ai cittadini che occorre sacrificarsi per un bene superiore, che poi altro non è che quello dei mercati finanziari confronti dei risparmiatori o alla legge a favore delle multinazionali farmaceutiche) e della ricchezza di poche persone a discapito del popolo, che ormai non può più far figli, curarsi, permettere ai propri figli di studiare e, soprattutto, andare in pensione a un'età Non posso che votare contro questa legge elettorale, che corrisponde agli interessi di pochi. Non ci devono essere liste bloccate; ci si deve esprimere con voto

che sia frutto di una compagine omogenea di un programma di coalizione. Avevamo chiesto le preferenze e un premio di maggioranza, perché concepiamo la politica come servizio ai cittadini. Crediamo nel merito Crediamo nel merito che si guadagna sul campo e non perché si è proni alle segreterie di partito. Avremmo desiderato che i nostri parlamentari fossero scelti dagli elettori. Per questi motivi e tanti altri, che per questioni di tempo non riesco ad illustrare, Fratelli d'Italia vota convintamente no ad una legge che, di fatto, considera il voto del suo popolo carta straccia. Noi restiamo ancora convinti che le leggi elettorali si fanno per l'interesse dei cittadini e non per i partiti, per gli elettori e non per gli eletti. perché così oggi si sentono i cittadini italiani: sentono di non avere la possibilità di esprimersi. Quindi, ha ragione nel darmi pochi secondi. È ingiusto non aver prodotto una legge, che si poteva

che avere una legge è necessario, ancora più indispensabile è avere una legge giusta per una giusta democrazia. Oggi il cittadino non si esprime e pertanto io, in rappresentanza di questo - signor Presidente, la presunzione di sentirmi un cittadino della strada come mi vanto di essere - non parteciperò al voto perché non mi sento rappresentato.

2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938.

la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della sessione di bilancio. In relazione ai tempi di trasmissione del disegno di legge di bilancio, il Presidente renderà le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 126, 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del provvedimento martedì 31 ottobre alle ore 17. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. La settimana dal 6 al 10 novembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni sul disegno di legge di bilancio e sul decreto-legge n. 148 in materia finanziaria, presentato al Senato. La discussione di quest'ultimo provvedimento avrà luogo nelle sedute uniche, senza orario di chiusura, di mercoledì 15, giovedì 16 e, se necessario, venerdì 17 novembre, con inizio alle ore 9,30. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti sul disegno di legge di bilancio alla 5a Commissione permanente entro la mattina di mercoledì 8 novembre. La Commissione bilancio riferirà all'Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre. Per l'esame del provvedimento, il calendario prevede sedute uniche senza orario di chiusura fino a sabato 25 novembre, se necessario. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 18 di lunedì 20 novembre. Infine, su richiesta del Presidente del Gruppo del Partito Democratico, il Consiglio di Presidenza è convocato alle ore 15 di martedì 31 ottobre per valutare quanto avvenuto in Aula nel corso della discussione sulla riforma elettorale. Presidente, come già anticipato nella Conferenza dei Capigruppo, sottolineo che qui si dà per scontato un calendario basato su un disegno virtuale, perché ad oggi un disegno di legge di bilancio non c'è, ma già si inserisce in calendario. È ormai troppo evidente per gli italiani che qui i tempi sono stati dosati

come ha riconosciuto persino il senatore a vita Giorgio Napolitano; e ora stabilendo che necessariamente si inizierà la sessione di bilancio martedì su un testo che ancora non è pervenuto.

Le richieste sono due: dare la possibilità alla Commissione bilancio di esaminare i provvedimenti uno dopo l'altro;

lei ha anticipato che ci sarebbero state possibilità in relazione a eventuali novità pervenute dal Governo sulla legge di bilancio. Chiedo allora di fare altrettanto. Come si è detto di lavorare sulla legge elettorale

richiesta del senatore Endrizzi di variazione del calendario, nel senso di ritardare la

per determinare il calendario relativo ai lavori della legge di bilancio. Ritengo che qualsiasi altra proposta sia inammissibile la Conferenza dei Capigruppo era stata convocata per un determinato obiettivo e, se avessimo dovuto discutere altre questioni, sarebbe stata convocata con altro ordine del giorno. Credo che vada seguita una regola

una nuova finestra"), presentata al ministro Fedeli, per un caso di odiosa discriminazione nei confronti di ragazzi italiani e di ragazzi extracomunitari. Mentre il Ministro dello sport giustamente ha consentito ai ragazzi extracomunitari, iscritti a società sportive, di partecipare ai campionati nei loro settori di partecipazione, viceversa il MIUR ha impedito la partecipazione di ragazzi, iscritti a una scuola privata legalmente riconosciuta, la San Paolo di Parma, ai campionati studenteschi.

non c'è alcun onere per lo Stato, perché i ragazzi e gli accompagnatori di questa scuola pagano di tasca loro la partecipazione. Chiedo allora che il Ministro

la partecipazione insieme ai colleghi ai campionati studenteschi, che sono un grande momento di partecipazione ed esaltazione dei princìpi dello sport. Chiedo pertanto che il Ministro dia una risposta sollecita alla mia interpellanza, naturalmente auspicando che questa odiosa discriminazione venga rimossa.

occupando i teleschermi e le pagine dei giornali, e che sono ben lontane dai problemi dei cittadini, ricevevo sulla mia casella *e-mail* la busta paga

che in Italia si vede tagliato a metà il proprio stipendio, tra tasse e tutto il resto. Il costo del lavoro, la difficoltà per le imprese di stare sul mercato, le difficoltà per i lavoratori di andare avanti con uno stipendio che non gli consente nemmeno di mantenere una famiglia. Questi sono i punti su cui vogliamo che il Governo si attivi e questi sono gli impegni che chiediamo al Governo per la prossima legge di bilancio, altrimenti ancora una volta avrete parlato di cose che al Paese non interessano.